ha risentito di una critica di fondo, da cui vorrei muovere per fare qualche breve riflessione. Questo Governo e questa maggioranza, nonostante la capacità che hanno mostrato in questo primo anno e mezzo di legislatura la capacità di tenere la rotta in una tempesta finanziaria che minacciava impatti ben più drammatici sul piano dell'economia reale e sul piano sociale, la capacità di dispiegare interventi che hanno saputo reggere l'urto di una crisi e salvare la coesione sociale del Paese, in un quadro di finanza pubblica che, data la condizione di partenza, non andava ulteriormente degradato (così come non è stato degradato) -, nonostante questa capacità di tenere in un momento tempestoso ed insicuro, nonostante questa prova di rigore e anche di efficacia,

ammettono che la crisi è alle spalle e, soprattutto, che questo Paese nel suo insieme ha saputo affrontarla senza disperdere il suo potenziale creativo e produttivo, per stare dentro, con le sue potenzialità espansive, alla ripresa che prende corpo. E l'attuale scenario non era del tutto scontato. Dobbiamo ricordare a noi stessi che non solo sono state avviate misure anticrisi adeguate per salvare l'apparato produttivo, quello creditizio e, da ultimo, le competenze professionali di questo Paese, ma, contestualmente, sono state varate azioni di riforma strutturali che hanno l'ambizione di cambiare profondamente il contesto entro cui si muovono i fattori di crescita del nostro Paese. Mi riferisco alla riforma della pubblica amministrazione, con la sua promessa di snellimento, di alleggerimento e di risparmio conseguente, al federalismo fiscale, con i decreti che stanno per vedere la luce e che dovranno riscrivere un nuovo patto fiscale fra Stato, cittadini e poteri locali, improntato all'efficacia delle prestazioni e alla responsabilizzazione dei centri di spesa, alla riforma dell'università e delle scuole, che ha ormai preso il via per essere una leva fondamentale per la coesione morale e la crescita intellettuale della nostra comunità nazionale. A questo si aggiunge la stessa riforma della legge sulla contabilità dello Stato (legge di stabilità), che, attraverso meccanismi più trasparenti, si fa carico di assumersi la questione delle questioni, quella del debito pubblico, con l'obiettivo di controllarlo attraverso una pervasiva e sistematica azione dello dello Stato di valutazione della spesa nei diversi centri di impiego e del loro impatto in termini di risultati. Proprio la riduzione della spesa e la sua qualificazione ci sembrano il vero spazio in cui gli spiriti riformatori devono dare testimonianza concreta di coerenza, sconfiggendo quel partito della spesa che in questi anni ha avuto il sopravvento con il lascito che oggi dobbiamo amministrare per non compromettere il futuro delle nuove generazioni. Sono certo, signora Presidente e colleghi, che questo spirito riformatore troverà ancora il tempo e il modo di esprimersi, come già accaduto in diverse occasioni in questa legislatura, con la concretezza e la determinazione

Signora Presidente, credo di aver già anticipato nella mia relazione di apertura le risposte da dare ai pochi, ma assolutamente significativi interventi dei colleghi in discussione generale. Posso solo rapidamente ripetermi in parte e comunque riconfermare,

e, se parte degli interventi dell'opposizione - in particolare del collega Morando - sono in gran parte condivisibili sulle proposte, lo sono ovviamente meno in ordine al giudizio totalmente negativo su questo testo, se non altro perché in non poche delle modifiche introdotte alla Camera il Governo ha risposto esattamente a molti emendamenti presentati qui in prima lettura, anche dal centrosinistra. Ecco perché la cautela (chiamata dall'opposizione mancanza di coraggio) che il Governo ha mantenuto fino a d'oggi, soprattutto per il rigore dei conti su alcune proposte condivise tra centrodestra e centrosinistra, deve vederci disposti a insistere affinché negli imminenti interventi legislativi

occorre anche agire contro il contingentamento del credito, fondamentale per la ripresa delle imprese, e insistere altresì sul monitoraggio attento che il Governo già attua sulla piaga dei pagamenti della pubblica amministrazione.

finanze*. Signora Presidente, ringrazio i relatori di maggioranza e di minoranza e tutti gli intervenuti a questo dibattito concentrato. concentrato. Ovviamente condivido quanto testé detto dal relatore Saia, e cioè che allo stato attuale la finanziaria non è modificabile. Ma non è modificabile non solo per una questione di carattere formale, perché ormai siamo in terza lettura, ma anche perché la sua struttura è difficilmente pensabile in un modo diverso. Abbiamo cercato, con l'attuale manovra, di tenere ferma la barra

per certi aspetti, incoraggiante perché, se guardiamo ad esempio alla crescita del debito pubblico che c'è stata da noi, vediamo che essa è inferiore rispetto a quella che si è realizzata nel corso del 2009 in altri Paesi europei ed extraeuropei. quello che - anche senza troppi interventi pubblici - ci ha consentito di superare questa fase e di guardare con ragionevole ottimismo al futuro è proprio il fatto che la spesa pubblica è stata tenuta molto stretta. Non basta tenere stretta la spesa pubblica, ovviamente, ma bisogna anche guardare avanti per cercare di affrontare con possibilità di successo le occasioni che ci deriveranno da una possibile ripresa dell'economia, dotare il Paese delle necessarie riforme strutturali che consentiranno, appunto, di ottenere questo obiettivo. Molte di queste riforme, però (basti pensare alla scuola, all'università, alla pubblica amministrazione, alla giustizia civile, in modo da avere processi civili più rapidi, - perché no? - anche alla riforma della legge di contabilità), sono già state realizzate. Ovviamente necessitano di essere implementate, ma il cantiere delle riforme è assolutamente aperto e *in progress*. A tutti piacerebbe poter ridurre in maniera consistente l'imposizione fiscale ed offrire più *chance* a tutti i cittadini, ma bisogna tener presente che in momenti di difficoltà economica non sempre ciò è facile e ottenibile. Per diminuire la pressione fiscale, infatti, in qualche modo bisogna diminuire consistentemente la spesa pubblica: mi domando se ciò si possa fare in E, d'altronde, non si può non ringraziare il Parlamento per essersi reso conto in questa circostanza come sia inopportuno accelerare sulla strada della spesa pubblica, perché essa comporta - magari non immediatamente, ma in un prossimo futuro - un aumento della pressione fiscale, se non è compensata compensata da altre diminuzioni corrispondenti. E aumentare la pressione fiscale non vuol dire altro che gravare sugli strati più deboli della popolazione, quelli che possono difendersi

il Parlamento non trova la ragione della propria democraticità nell'aumento della spesa, ma nella tutela dei più deboli, che sono i contribuenti più esposti all'aumento della pressione fiscale e meno in grado di difendersi. In sostanza, nel Parlamento si trova la forza del Paese, che è quella di contrastare le *lobby* (piccole e grandi: non sono solo i grandi gruppi d'interesse, ma i gruppi diffusi di

siccome questa è l'ultima occasione in cui il Parlamento italiano approva una legge finanziaria, mi lasci

nei momenti in cui occorreva fare manovre per entrare nella moneta unica e quando si sono dilapidati i tesoretti. Il Paese in questi anni è cambiato, soprattutto perché è cambiato il sistema politico: siamo passati da un sistema un sistema proporzionale ad uno sostanzialmente bipolare; è cambiato il quadro economico, non solo italiano ma mondiale; si sono aperti i mercati e ha preso avvio la globalizzazione: è ovvio che anche il modo di fare le leggi finanziarie non poteva restare lo stesso del passato. finanziaria era uno strumento disegnato per un meccanismo proporzionale, che oggi non esiste più: siamo passati da un'affermazione della centralità del Parlamento alla necessità di arrivare a decisioni più rapide per far fronte soprattutto alla maggiore alla maggiore velocità di reazione dei mercati e dei sistemi economici internazionali, tra loro così correlati. È questa quindi l'occasione per dire addio senza rimpianti alla vecchia legge finanziaria, non senza ricordare, però, chi da 31 anni l'ha accompagnata: dai protagonisti che l'hanno ideata e gestita alle più semplici storie personali di tanti dei quali la legge finanziaria ha segnato, con il ritmo immutabile delle stagioni, il trascorrere dell'esperienza umana.

si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato 1791-B

Si tratta di una giornata particolare: vi sono esigenze di armonizzazione dei tempi e di definizione dei lavori entro tempi contenuti che consentano anche ai colleghi di raggiungere le proprie sedi, date le difficoltà oggettive che si vivono in queste ore per muoversi all'interno del Paese a causa del maltempo.

è risuonata la volontà di porre mano ad un settore così delicato e in grande sofferenza: ve ne è traccia, peraltro, anche nella prima stesura del disegno di legge finanziaria in alcuni emendamenti che la maggioranza medesima ha presentato, salvo poi fare clamorosamente retromarcia, tornare indietro, modificare l'atteggiamento e, di fatto, costringere l'ambito della Difesa a una condizione di vita stentorea e comunque inadeguata. Questo emendamento punta ad una rivalutazione del comparto, ad un'implementazione delle risorse finanziarie, e a questo fine propone, nei termini indicati dall'emendamento medesimo, il recupero di significativi finanziamenti.

nel senso di prevedere detrazioni o l'attribuzione di un assegno, cioè il meccanismo dell'imposta negativa, per i redditi medio-bassi. Segnalo, in particolare, la parte dell'emendamento che si riferisce alla proposta di ridurre significativamente la pressione fiscale sul lavoro femminile. Siamo un Paese nel quale la partecipazione delle donne alle forze di lavoro è particolarmente bassa. Se si dovesse indicare qual è il principale fattore produttivo non utilizzato dal nostro sistema economico, certamente si dovrebbe concludere che questo fattore è costituito dalla presenza nel nostro Paese, in particolare nelle aree dell'obiettivo 1, di una quantità enorme di giovani donne in età di lavoro, che hanno una formazione migliore di quella dei coetanei maschi e che hanno una disponibilità all'impegno e al sacrificio anche maggiore di quella dei coetanei maschi, ma sono talmente sfiduciate circa la possibilità di trovare un impiego non scendono sul mercato del lavoro, così tenendo bassissima la partecipazione alle forze di lavoro. Queste disponibilità, queste forze, cioè, non compaiono nemmeno negli indici dell'occupazione e della disoccupazione. proposta è molto precisa e puntuale: creare una situazione, attraverso un'iniziativa di sperequazione favorevole alle donne, tale per cui un'impresa che dia lavoro ad una donna a parità di salario, a parità di prestazione, a parità di produttività debba far fronte ad un costo inferiore e creare una situazione in base alla quale all'interno della famiglia il lavoro femminile non sia penalizzato, in termini di rendimento e di reddito, rispetto al lavoro maschile. Soltanto attraverso questa misura noi potremo progressivamente determinare una situazione nella quale questa grande risorsa al servizio dello sviluppo del Paese potrà essere effettivamente utilizzata. Faccio notare, in particolare al rappresentante del Governo, che continua a dire che proponiamo emendamenti coperti con aumenti di pressione fiscale, che questa parte dell'emendamento potrebbe essere tranquillamente coperta dall'ultima parte dell'emendamento stesso, cioè l'articolo 2-*bis,* dove si propone di ridurre la spesa corrente primaria nell'entità necessaria per finanziare questo intervento di riduzione della pressione fiscale sul lavoro

uscire dalla recessione durissima che abbiamo attraversato per iniziare a camminare con un ritmo più elevato di quello che,

Presidente, illustro gli emendamenti 2.23, relativo al Patto di stabilità interno per 2.71, con il quale si chiede la soppressione dei commi dal 183 al 188 dell'articolo 2 che introducono una modifica rilevante all'ordinamento degli enti locali. Il complesso delle norme previste in finanziaria agli enti locali hanno prodotto la decisione da parte dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani di interrompere le relazioni istituzionali con il Governo. Il 10 dicembre scorso davanti a Montecitorio si è tenuta un'assemblea straordinaria del consiglio nazionale dell'ANCI, con la presenza di sindaci di tutti gli schieramenti politici, che ha votato un ordine del giorno con il quale si stigmatizza duramente la presenza in finanziaria di norme relative all'ordinamento degli enti locali e la totale assenza di modifiche del Patto di stabilità interno. L'unico elemento positivo contenuto nella finanziaria che ci viene proposta, e che anche noi come Gruppo del Partito Democratico riconosciamo, è la restituzione di ciò che è dovuto ai Comuni per quanto riguarda l'ICI sull'abitazione principale a partire dall'anno 2009 anche se, purtroppo, mancano ancora 350 milioni di euro per l'anno 2008.

che si accompagna e si sovrappone alla situazione di drammatica crisi economica che i lavoratori e le imprese stanno subendo in queste settimane. Si è poi voluta introdurre una norma relativa all'ordinamento degli enti locali che è del tutto illegittima per quanto riguarda lo strumento della legge finanziaria anche alla luce delle nuove norme di contabilità che abbiamo approvato. Certamente una riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori era possibile ed era già contemplata nel patto siglato tra associazioni delle autonomie e Governo nel 2007. Il punto è che qui la si è voluta fare attraverso la norma della legge finanziaria, in modo demagogico per sostenere che i costi della politica sono tutti a carico degli enti locali, quando invece è vero il contrario.

molto penalizzati per quanto riguarda le regole di questo Patto di stabilità interno. In più si arriva al paradosso che con queste norme si aboliscono da subito tutti gli organi circoscrizionali in tutte le città italiane, senza fare differenza tra le grandi città, le aree metropolitane - dove vi sono vere e proprie municipalità che hanno compiti di servizio dei cittadini - e tutti gli altri Comuni. Si arriva all'assurdo che il Comune di Venezia, che voterà nel marzo di quest'anno, non potrà istituire le municipalità, e si abolisce ovunque il direttore generale, generale, figura introdotta all'inizio degli anni '90 proprio per dare managerialità ai Comuni e per mettere sotto controllo la spesa. Con queste norme andate nella direzione opposta al federalismo qualunque sia la finanziaria che uscirà da questo Parlamento, sia chiaro che l'atteggiamento di protesta molto forte in Italia assunto dai Comuni italiani costringerà questo Governo e questa maggioranza a modifiche che noi del PD sosterremo.

Si tratta di un emendamento che affronta un tema molto discusso, soprattutto nel passaggio in prima lettura qui al Senato. Si riferisce alla cedolare secca, all'introduzione cioè di un'imposta che permetta di avere una tassazione pari al 20 per cento del canone di locazione per i proprietari e che consenta contestualmente al soggetto che affitta l'immobile di dedurre una parte dell'affitto che paga fino ad un massimo di 3.000 euro. È una misura razionale, intelligente, utile. C'eravamo fatti la speranza durante la discussione nella prima tornata sulla finanziaria al Senato che finalmente questa misura potesse vedere la luce, potesse vedere la luce, contribuendo a segnare con un profilo di qualità e di innovazione i contenuti di questa finanziaria. Non è stato così. Ci si è limitati al recepimento di un ordine del giorno da parte del Governo. Il problema è rimasto aperto a dimostrazione che il tema ha una sua forza e motivazione assolutamente fondata perché questa è una misura che potrebbe generare una emersione del sommerso in termini davvero rilevantissimi; è una misura che si paga da sé, perché per il primo anno costa, ovviamente in termini di riduzione del gettito preventivabile, circa un miliardo, ma è una misura che già dal terzo anno va in pareggio e potrebbe cominciare a generare utili per l'erario. Ovviamente si tratta di lavorare su un modo di affrontare le problematiche fiscali in cui si determina una convergenza di interessi

delle norme sui contratti che regolano il settore questa quota traendone un beneficio. Tutto questo sarebbe utilissimo. Abbiamo già avuto esperienze, ad esempio con l'introduzione della misura dello scomputo del 36 per cento sulla ristrutturazione edilizia, che hanno dimostrato come dalla convergenza di interessi emerga un volume potenziale di ulteriori risorse anche per l'erario. La fondatezza di questa impostazione è dettata dal fatto che il Governo e la maggioranza alla Camera hanno ritenuto di introdurre in via sperimentale tale misura per il territorio dell'Aquila, ma ovviamente è un pannicello caldo. Potrà servire in quella situazione, ma di fatto non sposta niente in termini di efficacia

introdurre nella nostra legislazione. Tra l'altro, voglio ricordare al rappresentante del Governo, il vice ministro Vegas, che se c'era un modo per dare un senso all'utilizzo delle risorse rivenienti dallo scudo fiscale era quello di usare un'entrata *una tantum* in modo appropriato per finanziare l'innesco, uno *start up*, di una misura che avrebbe potuto generare poi benefici di carattere strutturale. Noi sappiamo che ammontano a milioni le case che risultano non utilizzate, mentre poi è noto che in buona parte in qualche modo sono utilizzate nei

l'esigenza, in questo Paese, di prevedere interventi che efficacemente, utilmente e con soddisfazione dei soggetti interessati e coinvolti potessero aiutare meccanismi e dinamiche di contrasto all'evasione e all'elusione. Questa è una misura esemplare. Non attuarla è sicuramente una penalizzazione per quei cittadini interessati, è un danno per il rilancio dell'economia del sistema Paese e, soprattutto, è un'ulteriore perdita di occasione per compiere un'operazione più equa e giusta sul piano della fiscalità generale.

oggi incombe sulla ripresa economica in atto è rappresentata dalle difficoltà di finanziamento delle scelte di spesa delle famiglie e delle imprese. Nel nostro Paese questa difficoltà di finanziamento delle scelte di spesa delle imprese è aggravata dal fatto che la pubblica amministrazione, che ha dei debiti nei confronti delle imprese stesse, nel corso di questi ultimi mesi è andata aggravando i tempi di pagamento, cioè i tempi di pagamento della pubblica amministrazione si stanno allungando. che la spesa pubblica ha nel determinare il volume complessivo della spesa per investimenti e per consumi, ciò aggrava il *credit crunch*, cioè il contingentamento del credito nei confronti delle imprese, mettendo spesso le imprese in condizioni tali da dover assumere provvedimenti di riduzione dell'occupazione e fare gravi scelte sul versante della rinuncia a collaboratori atipici che lavorano all'interno dell'impresa a causa delle difficoltà di finanziamento che si aggiungono, per i ritardi della pubblica amministrazione nei pagamenti, alle difficoltà di accesso al credito che riguardano il rapporto tra imprese e banche. In coerenza con un punto fondamentale del programma del Partito Democratico, quello con il quale ci siamo presentati alle elezioni, avanziamo una proposta precisa che riguarda la scelta di eliminare situazione con un intervento organizzato attorno al ruolo della Cassa depositi e prestiti, certamente oneroso nell'immediato per il bilancio dello Stato. Questo intervento Stato. Questo intervento sarebbe tale per cui le imprese cedono il credito alla Cassa depositi e prestiti da cui vengono pagate ed è poi la Cassa depositi e prestiti, attraverso un complesso di operazioni finanziarie, a rivalersi nei confronti delle amministrazioni colpevoli di ritardato pagamento. Il Governo, attraverso l'assestamento, ha compiuto scelte che vanno in questa stessa direzione ma è del tutto evidente che esse sono al di sotto delle esigenze. Noi proponiamo attraverso l'emendamento 2.12 di fare un salto di qualità su questo versante; si tratta, ripeto, di una delle questioni più rilevanti al fine di accelerare il ritmo della ripresa nel nostro Paese.

2.13 torniamo a porre con forza il tema dello sviluppo produttivo nel nostro Paese, delle politiche industriali e degli strumenti a sostegno degli investimenti delle imprese. Torniamo inoltre a riproporre con forza procedure automatiche trasparenti immediatamente esigibili per le imprese la riattivazione del credito di imposta per gli investimenti, non solo per la ricerca ma anche nelle aree sottoutilizzate. È grave che non si voglia mettere in campo uno strumento di incentivazione proprio in questo momento nel quale la crisi ha messo in evidenza tutte

capacità di trasferire nei processi produttivi le innovazioni che anche il mondo della ricerca pubblica e privata è riuscita a produrre nel nostro Paese. Questa finanziaria affida un po' di risorse al CNR e all'ENEA perché animino lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie perché sostengano gli investimenti delle imprese in direzione del recupero di una nuova capacità competitiva negli scenari produttivi e di mercato che oggi si vanno configurando. Ma quelle risorse risulteranno non correttamente impiegate se mancano strumenti per garantire il flusso degli investimenti necessari per rilanciare l'economia e gli assetti produttivi del nostro Paese nel quadro di nuove politiche industriali che sappiano assumere le priorità che a livello mondiale oggi i Paesi più accorti assumono, e cioè i temi della sostenibilità ambientale e di come l'innovazione nei cicli produttivi e nella qualificazione dei prodotti può garantire un risultato significativo anche sul versante del consumo delle materie

deve rispondere in merito alla scelta del Governo di respingere le proposte che nel corso della discussione della sessione di bilancio l'opposizione del Partito Democratico ha avanzato, l'argomento che non sarebbero disponibili in questo momento le risorse necessarie in condizione di equilibrio di bilancio, cioè mantenendo la stabilità della nostra finanza pubblica. In qualche caso si è spinto a dire che sarebbe bello, ma non si può;

Il tipo di proposte che avanziamo è ben rappresentato da questo emendamento 2.14, nel quale avanziamo la seguente precisa c'è una legge delega dello Stato perfettamente in vigore, approvata in particolare in quest'Aula con un concorso molto ampio, tant'è che viene definita legge Brunetta, ma più correttamente dovrebbe essere chiamata legge Brunetta-Ichino, perché alla definizione da quella riforma certamente il Gruppo del Partito Democratico e, in particolare, il professor Ichino hanno dato un contributo rilevantissimo. Avanziamo dunque una proposta semplice: associamo associamo all'attuazione della legge Brunetta‑Ichino obiettivi di risparmio (amministrazione per amministrazione, ufficio per ufficio) e con quei risparmi costituiamo un fondo; in tanto ci saranno i risparmi, in quanto naturalmente l'attuazione della legge Brunetta andrà avanti con rapidità, e quindi, se ciò avverrà, i risparmi si costituiranno rapidamente.

cioè in particolare per eliminare progressivamente dalla base imponibile dell'IRAP il costo del lavoro, la cui presenza nella base imponibile dell'IRAP è elemento da tutti considerato particolarmente fase della crisi, ad una strategia di ripresa rapida dello sviluppo del nostro Paese. Signor Vice Ministro (mi rivolgo tramite lei al Ministro dell'economia), il Ministro dell'economia non può risponderci

ridurre la spesa corrente primaria non attraverso tagli, ma tramite un'azione di riforma della pubblica amministrazione e associando a quest'attività a quest'attività una di finanziamento della riduzione della pressione fiscale sul lavoro. La verità è La verità è che il Governo e la sua maggioranza non hanno la forza politica necessaria per assumere questo orientamento; la verità che proponiamo soluzioni onerose, perché questa non costa assolutamente niente: certo, lancia una sfida e determina una situazione completamente nuova. Qual è la difficoltà politica che abbiamo avuto a ridurre la spesa corrente primaria nel corso di tutti questi anni? Il fatto che non ci siano forze organizzate che premano nella società sulla politica per il conseguimento di quest'obiettivo. Se approvassimo un emendamento o soluzioni di questo tipo - su cui torneremo, certo, nello sviluppo del dibattito di politica economica, anche nei prossimi mesi

coloro che premono sulla politica non per ridurre la spesa corrente primaria, ma tendenzialmente per aumentarla a discapito delle prospettive di sviluppo del Paese. *(Applausi dal

in materia di efficienza termica degli edifici. Apprezziamo che il Governo abbia prorogato le agevolazioni del 36 per ristrutturazioni degli edifici e soprattutto che abbia stabilizzato la riduzione dell'IVA al 10 per cento. Riteniamo molto grave che non si proroghino invece gli interventi di efficienza termica degli edifici. Il fatto che a Copenaghen siano stati raggiunti risultati limitati non toglie che permangano comunque i limiti - accettati del resto dal Governo italiano posti in sede comunitaria. Certamente, la presenza di incentivazioni in questo campo costituisce uno strumento molto efficace per migliorare l'efficienza energetica del sistema Italia, ma per funzionare occorre che questi interventi agevolativi offrano un orizzonte sufficientemente stabile. Si tratta di investimenti per le famiglie non del tutto banali, dell'ordine di di alcune migliaia di euro - fino a 10.000-15.000 euro per un impianto fotovoltaico - e questo richiede la presenza di un orizzonte stabile. Quindi, lungi dall'eliminare questo intervento, si dovrebbe piuttosto renderlo stabile. Ricordo che con pochi euro si attiva una filiera molto importante che riguarda un settore produttivo ben presente nel nostro Paese, una fitta rete di installatori di impianti, una rete altrettanto cospicua di professionisti chiamati a progettare questi impianti e ad asseverarli dal punto di vista tecnico. Non si capisce, un intervento che con poco investimento produce un effetto così positivo per il sostegno dell'economia e per la qualità ambientale del nostro Paese non venga previsto dal Governo.

*(PD)*. Signor Presidente, vorrei richiamare con poche parole l'attenzione del Governo e dell'Aula sulle conseguenze di questa finanziaria sull'università e sulla ricerca. Il Governo non può non tenere conto delle parole di grande responsabilità che in questi mesi il mondo accademico e della ricerca, in particolare, i rettori delle università italiane, hanno adoperato

delle gravissime preoccupazioni che sono state sollevate dai rappresentanti del mondo accademico e della ricerca italiana sulle condizioni - definite drammatiche il mondo accademico e della ricerca italiana. È vero che la finanziaria che stiamo discutendo attribuisce alle università statali 400 milioni di euro a parziale reintegro - per il solo 2010 - del taglio di 678 milioni previsto dalla manovra dello scorso anno; peraltro, non prevede alcuna integrazione per gli atenei non statali. Con grande responsabilità la Conferenza dei rettori aveva indicato in 500 milioni - e non in 400 milioni per le università statali, e in almeno 50 milioni per le università non statali, il fabbisogno minimo complessivo per garantire il normale funzionamento delle università per l'anno 2010. Quindi deve essere chiaro che, senza fondi integrativi assegnati a breve termine e senza misure compensative, le condizioni di tutte le università italiane peggioreranno in modo significativo nella maggior parte dei casi, peggioreranno in modo irreversibile. Tutto ciò non ha a che fare con una normale razionalizzazione che sia volta a tagliare eventuali sprechi, pure riconosciuti presenti dai rappresentanti del mondo accademico nel funzionamento delle nostre università. è di grave impedimento per la programmazione del mondo accademico e della ricerca futuro, per il primo triennio, il fatto che non ci sia alcuna indicazione circa l'aumento del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011 e nessuna indicazione per le integrazioni dei finanziamenti per l'anno 2011. In queste condizioni di incertezza, moltissimi atenei non saranno in grado già nei prossimi mesi di svolgere alcuna programmazione. Questo stride con due provvedimenti, signora Presidente e cari colleghi, che sono stati presentati proprio nelle Aule parlamentari in questi giorni: la presentazione e l'inizio dell'*iter* parlamentare del disegno di legge di riforma dell'università, presentato dal ministro Gelmini e pure accolto con grande attenzione anche dal Partito Democratico, e contestualmente l'avvio delle attività dell'Agenzia nazionale dell'università e della ricerca, per la valutazione dell'università e della ricerca. Non si vede come, in queste condizioni economico-finanziarie, si possano appoggiare due provvedimenti che, al di là dei distinguo e delle discussioni, sono stati unanimemente apprezzati come grandi opportunità. Quindi, rischiano di essere vanificate pure le buone intenzioni che sono presenti in questi due importanti provvedimenti. un'ultima, ma forse la più drammatica, osservazione: le conseguenze di questa finanziaria e le conseguenze della mancanza di indicazioni e di integrazioni finanziarie per l'università e la ricerca per il 2011 manifestano quanto poco o nulla si stia facendo per garantire non solo la tenuta politica e gestionale del sistema nel corso del prossimo anno accademico,

solo fra un anno accademico, che potrebbero rendere impossibile per i prossimi anni l'ingresso di nuove generazioni di ricercatori nelle università italiane. Questa, per un Paese come il nostro, che vuol essere competitivo nella sfida di Lisbona e nella sfida della costruzione di una società della conoscenza, è veramente una resa che non ci possiamo permettere e che rischia di classificare irreversibilmente in serie B il nostro Paese.

Signora Presidente, nel rispetto della volontà di non impegnare eccessivamente l'Aula del Senato con numerosi emendamenti, insieme ad alcuni colleghi abbiamo raggruppato in un unico testo tutte le problematiche non risolte della questione che riguarda il terremoto dell'Abruzzo. un'operativa risposta a coloro che ritengono nel linguaggio mediatico di aver ragione avendo rivolto al Paese una generica informazione che più o meno dice: abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, anzi ci siamo rivolti a quel disastro, a quel sisma

Politicamente parlando, di fronte all'accusa rivolta da parte di alcuni colleghi, soprattutto della Lega, ma penso anche di altre parti rappresentate nella maggioranza, secondo cui per questo Abruzzo si sarebbe fatto molto e di più, provo ad elencare, in modo da rappresentare, così illustrandolo, questo emendamento, tutte le questioni su cui non è stato fatto nulla e nemmeno iniziato: ne abbiamo ampiamente dibattuto in Commissione bilancio, ma in quella sede il vice ministro Vegas, in rappresentanza del Governo, ha dato alla sua maggioranza un *input* abbastanza chiaro. Ebbene, signora Presidente, nulla togliendo all'emergenza, molto ben gestita dalla Protezione civile di uno Stato che ha il dovere di comportarsi in questo modo in qualunque parte del mondo, le segnalo che anche nella finanziaria non c'è alcun impegno economico-finanziario per la ripresa delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, agro-industriali, commerciali, artigianali,

Non c'è nulla per la ricostruzione e la riparazione dei palazzi storici. Non c'è nulla per la proroga delle indennità riconosciute ai collaboratori coordinati e continuativi: sono famiglie che lavorano, signora Presidente, e che a Natale non avranno nulla, non solo gli 800 euro che per alcuni mesi sono stati dati loro, ma non avranno nulla. Non c'è nulla per la zona franca urbana. Lei sa che, a valle di una famosa discussione in Commissione ambiente in fase di conversione in legge del decreto sul terremoto Abruzzo, riuscimmo ad inserire la zona franca urbana. Il Governo, però, con un *blitz* in Aula portò il finanziamento di quella misura a 45 milioni di euro per un intero quadriennio, ossia per gli esercizi dal 2009 al 2012, con ciò di fatto togliendo la possibilità che questa misura fosse effettivamente efficace. Non c'è nulla sul Patto di stabilità interno degli enti locali. Stiamo parlando, signora Presidente, di circa 8 Comuni nell'ambito di un cratere di una Provincia che ha bisogno di questa misura. Che cosa ha fatto il Governo con un *blitz* in finanziaria in prima lettura? Ha portato un emendamento del relatore nel quale ha riproposto questa misura per il solo Comune dell'Aquila. Peccato che nel decreto sul terremoto questa misura già vi fosse per il Comune dell'Aquila, signora Presidente. C'era per il 2009, e allora il Governo non ha fatto altro che estenderla al 2010, non aggiungendo niente di più di quanto ordinariamente un Governo dovrebbe fare. Non c'è nulla sugli indennizzi in favore dei Comuni della Provincia dell'Aquila per quanto riguarda le spese maggiori conseguenti agli eventi sismici e all'emergenza. Non c'è nulla sulle attività didattiche: la riforma Gelmini è stata applicata così come previsto, infischiandosene completamente della situazione di dramma ivi esistente. Non c'è nulla sul personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliare. Non c'è nulla sugli infortunati a causa del lavoro, per i cittadini rimasti invalidi in conseguenza degli eventi sismici. Infine, signora Presidente, non c'è nulla per gli straordinari di quel meraviglioso Corpo dei vigili del fuoco che tanto ha fatto e continua a fare In ultimo, ricordo ai colleghi - ve lo ricorderemo fino a che non ripristinerete questa misura che vi siete inventati una nuova ferrovia dall'Aquila a Tagliacozzo, che non serve a nessuno se non a chissà quale impresa, invece di ripristinare i fondi della Pescara-Roma che avete tolto con il primo decreto-legge.

dalla Protezione civile (questo Governo peraltro nulla ha fatto di più sulle tasse, in merito alle quali ai cittadini abruzzesi si chiede la restituzione per finanziare la ricostruzione, a differenza

tutto il Parlamento si sarebbe messo insieme, avrebbe con molta intelligenza individuato una tassa di scopo da utilizzare per quanto occorre fare. Invece continuate a dire che tutto è a posto, che tutto è in ordine; ma i fatti parlano chiaro, e soprattutto le cifre, che sono pari a zero, per gli argomenti ora indicati, parlano in maniera molto eloquente. *(PD)*. Intervengo per illustrare l'emendamento 2.54, soppressivo del comma 105 dell'articolo 2, comma che stabilizza l'utilizzo del TFR inoptato per finanziare spesa corrente. «Esprimo grande perplessità e preoccupazione per l'utilizzo delle risorse dei lavoratori a fini di spesa corrente»: non sono mie queste parole. Sono le parole di un collega del PdL, l'onorevole

ha pure respinto gli ordini del giorno con cui chiedevamo al Governo di informare puntualmente il Parlamento sulla consistenza dei fondi, sull'equilibrio tra il bilancio dello Stato e quello dell'INPS e, in sintesi, di garantire ai lavoratori la consistenza certa delle risorse di cui sono titolari. Le perplessità su questa scelta, infatti, sono molteplici. Non è chiaro, innanzitutto, se la quota di TFR destinata alla copertura della spesa corrente corrisponde effettivamente alla somma accertata a bilancio. Non è chiaro, quindi, se potranno continuare ad essere coperte le spese in conto capitale già previste dalla manovra finanziaria per il 2007 e non è certa, infine, la possibilità di restituire tutto il TFR ai lavoratori. Il suo utilizzo, poi, è sostanzialmente destinato alla copertura delle spese per il Patto per la salute e alla restituzione dell'ICI ai Comuni. Si finanzia, in questo modo, con il salario differito dei lavoratori, la spesa per la sanità e si ripristina la finanza locale, mutilata dall'improvvido intervento del Governo sull'ICI. Tutto questo non è solo finanziariamente opinabile, ma è anche, e soprattutto, socialmente irricevibile. I lavoratori che con questa crisi perdono reddito e lavoro sono chiamati a sostenere la finanza statale e a pagare ancora (oltre che con le imposte, che non calano perché nella finanziaria non c'è nessuna misura di defiscalizzazione e di alleggerimento del carico fiscale sul lavoro dipendente). In altri termini, la riduzione delle tasse di cui hanno usufruito in pochi, cioè coloro che il pagamento dell'ICI se lo sono potuto permettere, e, soprattutto, a sostenere il diritto universale alla salute che a tutti, *in primis* ai lavoratori, dovrebbe essere garantito.

fino a qualche settimana fa sembrava scontata: quella di non vendere i beni confiscati alla mafia. Nel Paese in questo momento c'è enorme preoccupazione: una legittima preoccupazione.

Nel 1996, con la legge n. 109, a seguito della raccolta di un milione di firme, grazie alla mobilitazione vitale del tessuto della società civile del Paese e grazie a "Libera", il Parlamento compì un'altra scelta:

sono in condizione di essere controllati e fanno parte di un mercato che può determinare legalità e sviluppo senza necessariamente l'intermediazione mafiosa, mentre escluse tassativamente la vendita dei beni immobili, dove, invece, l'intermediazione mafiosa attraverso i prestanome rischia di diventare l'elemento focale e fondamentale. Signora Presidente, nel Consiglio comunale di Corleone - così come

ma sapete benissimo che i comuni non hanno le risorse per poter comprare i beni immobili delle organizzazioni mafiose, le quali

Valgono poco le argomentazioni sui grandi successi nella lotta alla mafia, perché con questa scelta oggi Cosa nostra ottiene un grande risultato. Noi lo vogliamo impedire, diciamo in modo chiaro e netto che i beni non vanno venduti, e avanziamo la proposta dell'agenzia per la gestione dei beni confiscati alla mafia. Questa proposta, voluta dalla Commissione antimafia e dalla parte più moderna e attrezzata della società, oggi viene boicottata

Signora Presidente, illustro l'emendamento 2.58. Recentemente il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha ricordato, non per la prima volta, che nel nostro Paese ci sono circa 1,6 milioni lavoratori senza ammortizzatori sociali; 1,2 milioni sono lavoratori dipendenti circa 450.000 sono collaboratori. Per tutta risposta il ministro Sacconi ha dichiarato che la riforma degli ammortizzatori è rinviata a dopo le elezioni regionali. Non si capisce perché

collegato alla finanziaria, approvato recentemente in quest'Aula e in fase di approvazione definitiva alla Camera. Quindi non c'è bisogno, come sostiene sempre il Ministro, di una ulteriore legge delega in materia. Comunque, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, non è certo sufficiente, come prevede il maxiemendamento, l'incremento dal 20 al 30 per cento del 2008 delle indennità per i collaboratori monocommittenti. A questo riguardo vorrei ricordare, sono dati INPS, che nel che nel corso del 2009 su 10.000 domande presentate più di 8.000 sono state respinte e che solo 1.500 sono state accolte. Così come non è sufficiente la proroga della cassa integrazione in deroga. Noi insistiamo, le risorse ci sono. Anche in quest'Aula abbiamo più volte chiesto al Ministro una risposta al riguardo.

quindi, l'argomentazione che non ci sono risorse non può essere assolutamente sostenuta. Ecco perché noi insistiamo affinché con questo emendamento aggiuntivo si vari al più presto, quindi con la massima urgenza, la riforma degli ammortizzatori. Con il nostro emendamento noi proponiamo sostanzialmente tre interventi: in primo l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinati e per tutti i rapporti di lavoro a progetto. In secondo luogo, l'estensione della cassa integrazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato; infine, in via straordinaria per l'anno 2010 - in considerazione

della cassa integrazione da 52 a 104 settimane. Vorrei ricordare, anche a questo riguardo, che parliamo di fatti concreti, di numeri e di persone che versano in una condizione drammatica.

Signora Presidente, intervengo per illustrare due emendamenti, il 2.72 e il 2.78. Per quanto riguarda il primo, signora Presidente e colleghi, vale la pena di inquadrare, pur se brevemente, il problema, sottolineando la determinazione con la quale la maggioranza è pervenuta direttamente con la legge finanziaria allorché, saltando a pié pari ogni forma di confronto parlamentare, ha ritenuto di dover inserire l'istituzione o la costituzione di Difesa Servizi Spa. Parallelamente a Difesa Servizi Spa è stata anche promuova un'innovazione, che rappresenta l'espressione della genialità o della creatività del Tesoro, riguardante i fondi di investimento immobiliari. Che cosa succede? Succede che l'attacco concentrico finalizzato all'occupazione del potere - potremmo dire usando un lessico un po' arcaico rappresentato da tutta l'amministrazione della Difesa ha portato a determinare queste due creature che agiscono in simbiosi, che si integrano a vicenda, allo scopo non solo di gestire tutta la committenza, non solo di gestire tutto il patrimonio immobiliare, ma anche di pervenire, laddove dovesse rendersi necessario, alla sua alienazione. È interessante, almeno dal nostro punto di vista, osservare come vengano costruite le sinergie quando l'obiettivo è surrettizio: da una parte ci si diceva «state tranquilli, Difesa Servizi Spa non venderà il patrimonio immobiliare»; dall'altro, parallelamente, è stata determinata la costituzione di fondi immobiliari, che, per definizione, potranno vendere immobili. Quindi, potranno vendere caserme, potranno vendere caserme, poligoni: tutto ciò che dovessero ritenere, per l'appunto, alienabile, in quanto non indispensabile. Allora, ferma restando la gravità di questa decisione, che determinando una corsia preferenziale di fatto costituisce un pericolosissimo precedente all'interno della pubblica amministrazione, vi è da dire che, paradossalmente, il risultato di queste operazioni di fatto immobiliari, immobiliari, anziché consentire un'implementazione delle disponibilità finanziarie del settore della Difesa, di fatto le prosciuga solamente. alla Difesa andrebbero le noccioline. Per questo chiediamo che, riguardo alla valutazione patrimoniale originaria, venga riconosciuto almeno il 75

cioè, la sanatoria, ancorché parziale, del bilancio del Comune di Roma, che in questa battuta è stata valutata in 600 milioni, arriva grazie ad un'anticipazione di tesoreria invocata a valere su ciò che i fondi immobiliari determineranno con l'alienazione di caserme e quant'altro. Inoltre, benché in occasione del dibattito alla Camera (poi stroncato miseramente con la richiesta del voto di fiducia) la stessa maggioranza avesse chiesto che analogamente, quindi con la stessa procedura, venisse richiesta un'anticipazione di 510 milioni per le esigenze addestrative, logistiche e dell'area industriale della Difesa, per tale comparto non è disponibile un euro. Non ci si venga quindi a dire che le procedure non sono state stravolte; non ci si venga a dire che questo Governo è attento alle esigenze del comparto difesa e sicurezza, perché i fatti, i numeri, i riscontri oggettivi testimoniano il contrario. Non solo non si può procedere al reclutamento, all'addestramento, alle manutenzioni e a tutto ciò che ricade nella filiera di questo ambito della pubblica amministrazione, ma ciò che è della Difesa viene di fatto privatizzato e sottratto al controllo della stessa. Noi chiediamo che almeno il 75 per cento della porzione iniziale riguardo al valore assegnato dal demanio a ciascun bene venga riconosciuto alla Difesa. L'emendamento 2.78, signora Presidente e colleghi, riguarda l'altro ambito del comparto difesa e sicurezza, quello legato cioè alla Polizia di Stato, più in generale ai vari corpi di polizia. Noi chiediamo che, per sopperire a tutte le esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza, venga disposto il finanziamento di 300 milioni annui per gli esercizi 2010, 2011 e 2012; chiediamo inoltre che venga contestualmente autorizzata la stabilizzazione dei Vigili del fuoco discontinui, i quali, alla data della procedura selettiva, risultino

Noi sappiamo quanto *appeal* politico la maggioranza abbia esercitato a suo tempo, quando si è presentata al giudizio degli italiani; sappiamo che sul tema della sicurezza questa maggioranza e questo Governo hanno impostato gran parte della propria campagna elettorale, ottenendo anche, a mio avviso inopinatamente, straordinarie fortune. Ci pare che questo equivoco enorme, tragico debba essere chiarito una volta per tutte. Se davvero vi sta a cuore la difesa e la sicurezza di questo Paese, avete l'occasione giusta e buona per dimostrarlo

prevedendo un incremento e un ampliamento del cosiddetto contributo unificato, cioè della tassa sui processi. Il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo fino ad ora era dovuto nei processi civili e nel processo amministrativo, mentre ne risultavano esenti i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie. Con la previsione normativa che intendiamo sopprimere viene modificata la legge 2 aprile 1958, n. 319, che riguarda proprio l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi del lavoro del lavoro e, dunque, anche per queste controversie sul lavoro sarà dovuto il contributo unificato. Siamo di fronte ad un vero e proprio colpo di mano che cancella, di fatto, la gratuità del processo del lavoro e introduce una odiosa tassa che colpisce le fasce più esposte alla crisi. Si tratta, infatti, di una norma che ricadrà pressoché esclusivamente sui lavoratori, sui pensionati, sugli invalidi, sulle persone colpite da malattie professionali, persone che d'ora in poi dovranno pagare per poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Tutto ciò si manifesta mentre il Governo, al contrario, annuncia interventi in favore delle fasce più deboli e in un momento di profonda crisi economica momento di profonda crisi economica in cui, invece di aiutare i più deboli, il Governo decide di colpirli con un balzello odioso e vergognoso.

si richiede lo stanziamento, per la voce cooperazione e aiuto pubblico allo sviluppo, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

dato nelle assemblee, nei consessi, nelle occasioni di confronto internazionale alle quali ha partecipato e delle quali, naturalmente e legittimamente, si è vantato negli ultimi mesi.

immediate sulla nostra capacità di interlocuzione a livello internazionale con i Paesi in via di sviluppo, ma che contribuisce a minare la credibilità del nostro Paese, facendo venir meno la sua affidabilità, rendendo vane le parole spese e le parole date. In questa settimana vi sono pervenute richieste in questa direzione da gran parte del mondo dell'associazionismo, da gran parte di quel mondo che è impegnato sul terreno della solidarietà e che ritiene che, senza una politica di aiuto pubblico allo sviluppo che almeno mantenga i livelli

di comune accordo con la comunità internazionale, di portare allo 0,7 per cento del PIL il nostro impegno. Siamo invece regrediti dallo 0,22 allo 0,11 per cento che oggi, attraverso questa legge finanziaria e le risorse fino ad oggi, stanziate, noi registriamo. Per questo pensiamo che lo stanziamento lo stanziamento di queste risorse sia un atto dovuto del quale dovreste sentire la responsabilità e che chiediamo al Governo e alla maggioranza di considerare quindi con attenzione.

che ha a che fare con i tagli del Fondo per lo spettacolo ed evoca, sia pure implicitamente, il 2.39, che concerne il taglio di un altro settore contiguo, quello dell'editoria. La situazione è più grave ancora, signor Presidente, colleghe e colleghi (pregherei di riflettere su questo tema), di quanto sia stata nel momento in cui, nella precedente lettura, una discussione analoga avvenne anche in quest'Aula, ed è più grave perché le previsioni si sono rivelate persino al di sotto di quello che si supponeva solo tre-quattro mesi fa. Per di più, un recente decreto legislativo dell'ultimo Consiglio dei ministri in materia ha dato un colpo ferale all'obbligo di investire in film e audiovisivi italiani ed europei da parte delle emittenti televisive nazionali.

l'eliminazione del diritto soggettivo delle testate ad avere i finanziamenti dedicati all'editoria *non profit*, cooperativa, locale o di giornali per le minoranze di partito è un tassello di questa linea, che si conclude con altre due - permettetemi - chicche: da una parte l'annunciata cacciata dell'attuale consiglio, che tanto ha fatto, della Biennale di Venezia; dall'altra, ipotesi censorie sul *web*, la rete e la sua libertà. Insomma, signor Presidente, colleghe e colleghi, questi nostri emendamenti sono volti a ripristinare quella libertà di comunicazione, di cultura e d'informazione che purtroppo questo testo mette in discussione fortemente. Il vice ministro Vegas pronunciava ieri alcune parole troppo impegnative e discutibili sull'argomento della cultura quasi che la cultura, sia un bene secondario e voluttuario, una spesa inutile. No! Come dimostra uno studio dell'università di Torino, per un euro investito in cultura c'è un ritorno di cinque euro, per cui questi tagli sono anche masochistici rispetto al nostro Paese e ad uno dei suoi grandi beni e virtù. *(Applausi dal Gruppo

Mi limiterò a presentare quelle sulle tematiche del lavoro. Inizio dall'emendamento 2.6, che chiede la detassazione di una quota della tredicesima mensilità di retribuzione. Conosciamo bene, signor Presidente, la situazione di tutte le famiglie italiane, che non riescono più nemmeno ad arrivare alla terza settimana. Proponiamo quindi una detassazione di una quota pari al 15 per cento della tredicesima in modo da aumentare davvero il potere d'acquisto delle famiglie e da far ripartire così i consumi, e di conseguenza anche l'economia italiana. all'emendamento 2.55, relativo al TFR - già l'ho detto in discussione generale - non condividiamo affatto lo spostamento del TFR in bilancio. È un'operazione pericolosa, che creerà senz'altro debito pubblico; è un prestito forzoso che i lavoratori fanno allo Stato per coprire la spesa corrente senza che sia posto l'obbligo al Governo di rendere conto circa l'utilizzo effettivo delle risorse o i tempi di restituzione delle stesse. Quindi, con tale emendamento noi chiediamo la presentazione di una relazione trimestrale al Parlamento al fine di effettuare un monitoraggio relativamente all'utilizzo dei fondi del TFR per dar conto con dettaglio dei reali utilizzi delle somme e delle reali disponibilità dei fondi TFR esistenti, ripartite tra impegni di parte corrente e impegni in conto capitale, al fine anche di verificare la sussistenza dell'equilibrio contabile per quanto attiene ai flussi di entrata e di uscita aventi come riferimento il trattamento di fine rapporto. Con l'emendamento 2.59 2.59 chiediamo l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto o atipici. Si prevede che la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui alla legge n. 164 del 1975 e successive modificazioni, venga estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private. In pratica, si preferisce detto intervento a carattere universale invece di quanto stabilito al comma 130, che si limita ad ampliare i requisiti e la misura dell'istituto sperimentale di sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti.

l'emendamento 2.64 chiediamo di abrogare le disposizioni che reintroducono il cosiddetto *staff leasing*, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abrogando così la norma del Protocollo *welfare* del Governo Prodi, relativo alla legge n. 247 del 2007, con la quale si era provveduto a mettere fine a questa metodologia

di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, per un ammontare complessivo annuale non superiore ad un milione di euro. 2.8 riguarda l'IVA di cassa e propone di rendere permanente per i piccoli operatori economici il pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, modificando l'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 che prevede tale disposizione solo per un anno, aumentando il volume d'affari massimo per l'applicazione della norma da 200.000 a 300.000 euro. 2.29 chiediamo la soppressione del rifinanziamento della "legge mancia", inizialmente stabilito dal Senato in 50 milioni, e poi portato a 100 milioni dalla Camera, e provvediamo ad utilizzare tale somma di 100 milioni per incrementare il Fondo per le non autosufficienze.

Richiamo l'attenzione di tutti i colleghi su tale emendamento. presso i tribunali. Guardate che si tratta di una questione veramente molto importante. Ieri, lo dico senza spirito polemico, i poliziotti (definiti spregiativamente "panzoni" dal ministro Brunetta) si sono rifiutati di andare dal Ministro della funzione pubblica per un incontro sulla concertazione. Bisogna fare di più per la sicurezza, non solo a parole ma anche nei fatti. prevede una detrazione per carichi di famiglia. Si riducono i consumi intermedi delle amministrazioni centrali e i risparmi confluiscono in un fondo presso il Ministero

risorse per i confidi al fine di garantire i prestiti alle piccole e medie imprese "strozzate" dalle banche (lo sappiamo, lo diciamo e lo leggiamo sui giornali ogni giorno). Chiediamo quindi di incrementare le risorse per i fondi di garanzia ai crediti alle piccole e medie imprese ed agli artigiani.

non impegneremo tutto il tempo a nostra disposizione per illustrare i nostri emendamenti, perché siamo in terza lettura e credo che, al di là della circostanza che non sia stata posta la fiducia dal Governo la tempistica dei nostri lavori ci porti ad un esame del testo della finanziaria come se la fiducia fosse stata posta. Detto questo, è chiaro che che quelle che abbiamo sollevato sono questioni note e che abbiamo affrontato con i nostri emendamenti già in prima lettura. Esse riguardano il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali per i familiari e la famiglia in generale (che non trova nella finanziaria alcun tipo di tutela e di disciplina), l'allentamento del Patto di stabilità per i Comuni più virtuosi (per rimettere in circuito alcune risorse finalizzate agli investimenti e quindi alla crescita),

Ma c'è una questione sulla quale riteniamo sia opportuno e necessario soffermare la nostra attenzione, così come già hanno fatto altri colleghi dell'opposizione: quella dei beni confiscati. Non credo ci sia la necessità di fare qui particolari polemiche, però occorre sviluppare un ragionamento. Il Governo, qualche settimana fa, quando la polemica su questo tema aveva raggiunto toni abbastanza caldi, aveva annunciato che sarebbe intervenuto per ridisciplinare il meccanismo di confisca e di assegnazione dei beni con l'istituzione di un'agenzia dedicata. Questa Questa è una proposta che condividiamo, ma ci saremmo aspettati di trovarla già in finanziaria, nel maxiemendamento che alla Camera il Governo ha presentato e su cui è stata posta la fiducia. Di tutto ciò non vi è traccia in questo testo, se non per alcune norme che in qualche modo sono funzionali ad accelerare le procedure di assegnazione dei beni. Resta pertanto il vizio di origine, quello dell'incapacità strutturale dell'agenzia del Demanio di procedere alla gestione con la confisca e l'assegnazione, tant'è vero che anche la relazione che il commissario straordinario ha fatto sulla gestione dei beni confiscati - commissario che questo Governo vuole rimuovere, e non se ne capiscono, sinceramente, le ragioni, essendo una persona che ha ben operato in questo settore indica con esattezza che il vero problema riguarda il *gap* che c'è fra i beni che vengono confiscati e quelli che trovano una loro definitiva definitiva assegnazione. Tutto questo non si risolve tentando di fare cassa per la giustizia e per gli interni con la vendita dei beni confiscati, ma attribuendo ad un soggetto qualificato la possibilità di portare a compimento quest'operazione, che è strategica nel contrasto al crimine organizzato. Infatti, l'unica cosa che consente di avere strumenti efficaci di contrasto alla criminalità organizzata è colpire i patrimoni mafiosi. Voi però introducete norme, peraltro complesse e inutili, ad esempio con riguardo all'esercizio della prelazione da parte degli enti pubblici o delle cooperative composte da aderenti a forze armate o di polizia: o di polizia: questo sistema normativo serve solo ed esclusivamente come orpello a giustificare una procedura che è nefasta, perché consentirà certamente

ad un effetto negativo: solo ed esclusivamente, per che cosa? Per un'idea malsana, che è stata quella di immaginare di coprire le spese del fondo

di fatto è l'immediata alienabilità dei beni stessi. Ci saremmo aspettati che, almeno su questa norma, il Governo, presentando il maxiemendamento alla Camera, manifestasse un principio di ripensamento: invece, il testo tanto corposo, tanto corposo, quanto inutile che ci troviamo ad esaminare qua al Senato mette una pietra tombale sul contrasto ai patrimoni mafiosi a cui solo una nuova normativa, che abroghi quella che stiamo approvando ora, potrà porre rimedio. Questa è la ragione per cui quella al nostro esame è l'unica della norme che ci permettiamo di segnalare: nel contesto nel contesto del dibattito su una finanziaria che nulla dice di nuovo, non ha alcun sapore e alcun colore, se non quello di tentare di coprire con entrate *una tantum* spese correnti, l'unica cosa che appare in maniera emergente è questa normativa che viene utilizzata per far cassa, attraverso una partita di giro di risorse dei mafiosi, per chiudere alcune partite in sofferenza che riguardano l'impossibilità di garantire in maniera ordinaria le spese di funzionamento della giustizia e del Ministero dell'interno. Credo che queste siano le ragioni che dovrebbero quanto meno riportare ad un ripensamento su questa materia e a modificare qui al Senato il testo solo per questa parte: i colleghi della Camera non se ne avranno a male se rimanderemo loro la finanziaria rimettendo almeno in piedi uno dei pilastri della lotta alla criminalità organizzata. intervengo molto brevemente per sottolineare come al comma 52 si sia immaginato un meccanismo decisamente farraginoso rispetto alla vendita dei beni della mafia (definiamoli così); un meccanismo farraginoso anche nella tempistica e che crea dei problemi sia per il riacquisto - perché non mi pare che ci siano dei margini grandissimi di certezza che i terzi non appartengano una società ben individuabile - sia rispetto alla destinazione delle somme ricavate, le quali andrebbero, così come immaginato nel comma 52, al Fondo unico per la giustizia,

continuo a non comprendere, pur nella necessità che si ha di razionalizzare assolutamente le spese, perché il Ministero della giustizia debba continuare a spendere tanti danari

per gli stessi immobili. Oltretutto, arriverebbe ad una patrimonializzazione che sarebbe utile al Ministero della giustizia, laddove dovesse immaginare che il *leasing* possa andare in favore del Ministero o in favore eventualmente dei Comuni, laddove dovesse autorizzare a considerare il fitto come quota di *leasing* per l'acquisto degli immobili stessi. Lo dico perché è una questione, che peraltro ho affrontato e ancora sto affrontando come residuo della mia amministrazione comunale, che mi ha creato più di un problema, ma nella quale credo fermamente perché ritengo siano dei soldi buttati al vento, considerato che, in una piccola città come la mia, il Ministero spende oltre 2.600.000 euro per palazzi di giustizia che potrebbero ben essere acquistati a prezzo congruo, naturalmente con la valutazione giusta da parte del Ministero stesso. Peraltro, i Comuni hanno necessità e bisogno di utilizzare i beni confiscati per una serie di interventi nel sociale, interventi nel sociale, che con le nuove povertà diventano sempre più forti e importanti, quantitativamente e qualitativamente. I Comuni hanno bisogno di locali locali persino per gli uffici, perché sono costretti a pagare somme ingenti per sedi decentrate; hanno bisogno di immobili per le scuole, per gli asili, per i centri sociali per gli anziani, per i centri di aggregazione; hanno bisogno di locali per l'emergenza abitativa. Dall'altro lato, abbiamo dei fondi, delle ingenti somme del Programma che - lo dico da ex amministratore comunale - il più delle volte purtroppo vengono utilizzati in progetti che non lasciano assolutamente nulla sul territorio; progetti che passano per progetti di educazione alla legalità, ma che non lasciano traccia di sé sul territorio. Ricordo ancora dei progetti finanziati con 500.000 euro - che qualche volta per un'amministrazione comunale

tra i fondi che, ricordo a mente, dovrebbero essere 94 milioni di euro per il PON sicurezza, e quelli che possono essere i beni confiscati alla mafia, che ben possono essere utilizzati per gli scopi sociali che gli amministratori comunali chiedono a gran voce.

52. Ricordo una pagina cruda nell'occasione della mia attività professionale. Era la trattativa fra un mafioso e il proprietario di un bene ed era una pagina che dava delle risposte estremamente significative su ciò che è la criminalità organizzata. La trattativa era in questi termini:

se volete 150, io ve la pago 200». Quella persona non cedette alle richieste, anche se economicamente apprezzabili, e il 10 luglio 1991 venne uccisa. La mafia è questa! Sappiamo che colpire la mafia significa colpire i patrimoni mafiosi. Lo Stato ha operato una scelta etica dicendo che quei beni frutto del crimine devono tornare alla collettività. Su questo messaggio, profondamente simbolico e di grandissima valenza, oggi incombe l'opzione pragmatica, perché si vuole che qualora, nel termine massimo di 270 giorni, i beni confiscati ai mafiosi non vengano destinati a fini sociali, quei beni debbano essere venduti. Ciò significa che abbiamo assegnato una valenza meramente economica ad un'opzione fatta dallo Stato che era di espropriazione dei beni mafiosi e di assegnazione alla collettività. Il discorso va al di là del valore economico: è un problema di messaggi. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la relazione del commissario straordinario per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un organismo della Presidenza del Consiglio; è una relazione altamente positiva: il quadro sta cambiando, si lavora meglio, ottimi i risultati. Il ministro dell'interno, Maroni, ha annunciato di condividere la proposta che da più anni si avanza, quella della creazione di un'agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati. Allora, in un quadro che si sta sicuramente ottimizzando, che dà dei risultati positivi, perché oggi si vuole con una norma in un sistema che diventa positivo? Per quale motivo oggi dobbiamo lanciare da quest'Aula il segnale contrario all'alto segnale simbolico che lo Stato aveva dato in questi anni? Rafforziamo il sistema per l'assegnazione dei beni, ma non sottraiamoli alla collettività! Dobbiamo riaffermare questo principio. Non fate esclusivamente un discorso economico; andate oltre. Abbiamo bisogno anche di esempi e di messaggi forti al Paese! Sopprimiamo questo comma, che non porta utilità allo Stato e lo depotenzia di un messaggio forte che sta vedendo finalmente i risultati! Mi appello alla vostra coscienza, perché il nostro Paese ha bisogno di simboli, di messaggi, di parole chiare. La criminalità organizzata si combatte radicalmente e i suoi beni non sono beni qualunque: sono beni

essere contrario a tutti gli emendamenti

un piccolissimo segnale da parte del Governo in fase sperimentale sull'area della provincia dell'Aquila. Sono convinto che su questo tema ‑ ha ragione anche l'opposizione a sottolinearlo ‑ si possa innescare una serie di meccanismi e benefici positivi, non solo fiscalmente, ma anche sull'occupazione stessa, sulla possibilità di mobilità dei cittadini nel Paese e quindi la possibilità di Grazie.

lettura proprio un emendamento dell'opposizione a tal riguardo affinché fossero inseriti anche i prefetti nel controllo di detta vendita. Quindi, la farraginosità diventa anche un elemento

Grazie.

contrario a tutti gli emendamenti presentati, ovviamente con un invito generale al ritiro perché, se venissero ritirati, si supererebbe la contrarietà.

sia consentito, signor Presidente, di fornire semplicemente qualche chiarimento su alcuni dei problemi lumeggiati negli emendamenti, senza stare a ribadire il parere contrario su tutti. È chiaro che, in linea generale, piacerebbe a tutti aumentare le detrazioni fiscali, diminuire l'imposizione, aumentare la spesa e quant'altro ma, come qualsiasi famiglia, anche un Governo non può

stata sollevata l'opportunità di derogare al Patto di stabilità interno, ma quest'ultimo riguarda gli enti locali e lega tutto - enti locali, Regioni e Stato - al Patto di stabilità europeo, per cui deve esserci armonia tra i diversi livelli di governo.

Sulla questione della cedolare secca per gli immobili, è vero che l'ipotesi per la sola città dell'Aquila è riduttiva, ma permette di esaminare *in vitro* - quasi fosse un esperimento sociale - se il meccanismo funziona o no. ai pagamenti della pubblica amministrazione, lo ha già fatto presente il relatore, con l'assestamento abbiamo immesso 18 miliardi di euro per pagare i debiti. È chiaro che non si possono pagare tutti i debiti subito, perché altrimenti il deficit esploderebbe, ma una somma di tale entità, che serve anche agli enti locali,

è facile guardare ciò che non c'è, ma in realtà qui non si tratta di un bicchiere mezzo pieno, bensì di un bicchiere pieno a tre quarti, perché quello che è stato fatto per l'Abruzzo non è mai stato fatto per altre Regioni italiane: basti pensare alla ricostruzione integrale delle abitazioni. Per quanto attiene inoltre alla questione fiscale, le proroghe sono state

Devo contestare recisamente l'opinione che alcuni colleghi hanno sostenuto circa il fatto che la vendita dei beni sequestrati alla mafia sarebbe un favore reso a quest'ultima in realtà è un favore alla collettività e serve a mettere in

le risorse messe a disposizione sono, allo stato, sufficienti; speriamo di non impiegarle tutte se l'economia riprenderà moderatamente. Un'ultima osservazione al senatore Vita, che ha lamentato le carenze del Fondo per lo spettacolo.

*(PD)*. Signor Presidente, ancora adesso, in sede di formulazione del parere, il vice ministro Vegas ha intonato la solita cantilena: sarebbe bello, piacerebbe a tutti, ma...

non è tale da proporre al Governo il tema del reperimento di nuove risorse per far fronte agli interventi che noi proponiamo. L'emendamento 2.14 (l'ho già detto, ma lo voglio ripetere) è la dimostrazione fisica di quello che sto dicendo. Avete o no la forza politica, il coraggio, la determinazione necessari per assumervi un impegno di riduzione della spesa corrente primaria, applicando la riforma della pubblica amministrazione che è prevista dalla cosiddetta legge Brunetta? Se avete questa determinazione, noi con questo emendamento vi proponiamo di associare a quella iniziativa un risparmio di spesa e di utilizzarlo per diminuire progressivamente l'IRAP, riducendo la componente costo del lavoro dalla sua base imponibile. Non potete rispondere seriamente che non lo fate, che dite di no perché manca la copertura finanziaria, perché in questo caso non c'è bisogno di nessuna copertura finanziaria. Vi proponiamo di governare il Paese in modo diverso da come lo state facendo. Siete liberi di dire di no, ma non potete nascondervi dietro questo dito che ormai lascia scoperta la vostra mancanza di coraggio, di determinazione, di visione sul futuro del Paese.

qui in Senato, e anche alla Camera dei deputati, né il Governo né la maggioranza hanno mai dato alcuna motivazione per giustificare il rifiuto opposto a questo emendamento, che molto semplicemente chiede di rinnovare la possibilità per i cittadini di detrarre il 55 per cento delle spese sostenute per le ristrutturazioni dei loro immobili che abbiano conseguito un risparmio energetico,

persone, hanno fatto lavorare le imprese, hanno dato insomma ossigeno, soprattutto alle piccole imprese dell'edilizia. Se l'emendamento 2.15 non viene approvato, a partire dall'anno prossimo le famiglie italiane si ritroveranno nell'incertezza

lo strumento della detraibilità di una parte delle spese per le ristrutturazioni energetiche degli edifici sia un esempio simbolicamente molto importante, oltre che concretamente utile, di quell'intreccio virtuoso tra politiche ambientali e politiche economiche che in tutta Europa (e oggi non solo in Europa) è al centro degli sforzi dei Governi per fronteggiare gli effetti sociali ed economici della crisi e della recessione. Che il Governo italiano si muova in direzione opposta è la conferma della vostra incapacità, colleghi della maggioranza e rappresentanti del Governo, di immaginare per l'Italia una visione di sviluppo e di progresso che tenga insieme il benessere economico e l'interesse generale a vedere ridotta la bolletta energetica delle importazioni di greggio e a vedere conseguiti importanti vantaggi ambientali per tutti i cittadini. Questa è la ragione per cui con forza sosteniamo, e chiediamo al Senato di sostenere, questo emendamento

In prima fila alla mia destra vedo tre luci accese e due senatori

La risposta del Vice Ministro francamente è poco gradevole: non può essere che il bicchiere sia pieno a tre quarti. Il fatto è che questo Paese

una frase, sulle questioni di merito affrontate in questo emendamento. Se lo rilegga dopo le vacanze, ammesso che abbia tempo, e vedrà che il bicchiere è totalmente vuoto, e non pieno a tre quarti.

l'emendamento 2.31, soppressivo del comma 52 dell'articolo 2, interviene in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. L'articolo 2 del disegno di legge prevede che possano essere venduti immobili di cui non sia stata effettuata la destinazione entro i 90 giorni imposti dalla legge. La destinazione dei beni confiscati alla mafia è prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, che fu a suo tempo approvata all'unanimità dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato. Fino ad oggi si è sempre ritenuto assolutamente indispensabile mantenere l'asse portante della legge, che vieta la vendita dei beni confiscati e destina gli stessi ai Comuni, allo Stato, alla società civile, alle cooperative di giovani e di lavoratori. E questo veniva disposto per l'alto valore sociale, etico e politico riconosciuto unanimemente all'istituto in questione. All'inefficienza del procedimento di destinazione sociale dei beni il legislatore sembrava voler porre rimedio con il recente pacchetto sicurezza, approvato con legge n. 94 del 2009. Con il comma 20 dell'articolo 2 di tale legge, infatti, veniva previsto che la destinazione sociale doveva essere stabilita con provvedimento prefettizio nel termine complessivo di 180 giorni, prorogabile di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni complesse. Ora, dopo neanche tre mesi, senza che sia stato neppure possibile controllare i risultati della riforma voluta appunto tre mesi fa dalla maggioranza, il Governo smentisce se stesso prevedendo con questa norma che, se non si riesce a concludere il procedimento nei termini di cui all'articolo 2-*decies*, non si fa luogo alla destinazione sociale, ma si procede alla vendita del bene. Questa vostra norma ha generato fortissime e generalizzate critiche nella società civile e politica e critiche fortissime anche dalle associazioni contro la mafia (in particolare dall'associazione "Libera") e dalla stessa procura nazionale antimafia. Questa vostra modifica è gravida di responsabilità morale, prima ancora che politica, nel contrasto alla criminalità organizzata. Il Partito Democratico ha presentato in materia un disegno di legge per la lotta alla criminalità organizzata e la confisca e la gestione dei beni

beni (perfino il ministro dell'interno Maroni è intervenuto a sostegno della necessità di una tale agenzia). Ora voi con questa modifica vi prendete una grande responsabilità, perché in territori dove il potere condizionante della mafia e di tutte le criminalità organizzate è forte si può intuire facilmente chi potrà esercitare la facoltà di ricomprare i beni confiscati alla mafia, senza poi contare il danno che viene arrecato alle fasce deboli e quindi a tutta la società che virtuosamente usufruiva di questi beni confiscati alla mafia in termini di cessione per le emergenze abitative, per alloggi di famiglie, per cooperative di lavoro e giovani in territori di criminalità organizzata. Con questa norma, con questa vostra grave scelta voi indebolite la lotta alla criminalità organizzata e fate un favore alla

mafia, che il bene sequestrato appartiene alla collettività e che, invece, in questo modo lo si destina ad usi civili:

Ora, voi dite - e la prima osservazione è del senatore Li Gotti - che il bene appartiene alla collettività e quindi ne deve usufruire quest'ultima. Se il bene viene venduto, senatore Li Gotti, l'introito va alla collettività, va allo Stato, non è che venga restituito alla mafia;

Tra l'altro, la procedura con la quale si arriva alla dichiarazione definitiva della confisca da parte dell'autorità giudiziaria passa attraverso il sequestro e poi tre possibili ordini di ricorso. Se un ente vuole avvalersi del bene, può quindi abbondantemente prepararsi le pratiche da presentare

una volta che è stato definitivamente confiscato, e darlo a chi ne fa un uso sociale. Non vi è tutta questa complicazione, se si lavora con serietà;

finirà per essere riacquistato dalla criminalità. A parte il fatto che nelle procedure d'asta si può applicare regolarmente quanto previsto

sulla vendita di quel palazzo, se vi è il dubbio, si attirerà di nuovo il rischio che venga confiscato. Concludo dicendo che, in realtà, la procedura prevede prima di tutto che i beni vengano confiscati, e su questo il nostro Governo sta agendo meglio di tutti i precedenti. E non lo potete negare! *(Applausi

si può prevedere, dopo la confisca definitiva, di assegnarlo alla funzione sociale. Se non avviene questo, e non avviene o perché non c'è la richiesta di funzione sociale o perché c'è una cialtroneria da parte di chi deve procedere... allora si prevede che si dia con prelazione ai Comuni, quindi alla società, e alle cooperative delle forze di Polizia e delle Forze armate. Anche questo è un impiego di carattere sociale, e quando voi fate un emendamento che propone di abolire il comma 52 togliete alle cooperative delle forze di Polizia e delle Forze armate la possibilità di avvalersi di questo bene. Bel risultato sociale! Se poi alla fine non si riesce in tutto questo, allora lo si mette in vendita e i soldi verranno incamerati per la società nel bilancio dello Stato. dire che questo comma è un favore fatto alla criminalità o alla mafia mi lascia molto perplesso, lasciate che ve lo dica.

al presidente Ramponi, con tutta la cortesia che posso - che il senatore Garraffa si occupa di tali questioni da moltissimi anni: è un componente della Commissione antimafia, è siciliano di Palermo, ha sperimentato su di sé tante volte l'asprezza di un'opposizione alle organizzazioni criminali mafiose, e non è qui per fare piazzate, ma per parlare di cose serie. *(Applausi dal Gruppo* *PD).* Senatore Ramponi, che appartiene probabilmente al migliore dei mondi possibili: se noi ragionassimo di queste cose in Svizzera piuttosto che in Svezia, le cose che lei dice, che sembrano cose di assoluto buonsenso, avrebbero la forza del buonsenso. Purtroppo, nel contesto nel quale ci muoviamo, sono i sogni di un Peter Pan dell'antimafia, mi lasci usare questa espressione. Per la mafia, riconquistare il bene che le è stato sequestrato ha una forza e un valore simbolico di cui lei non può avere idea. Non è la questione esclusiva del bene materiale, del suo valore di mercato, non è l'affare, non è il *business*! È il fatto che in quella casa torna a comandare la mafia e non lo Stato! Il valore della legge che trasforma in ricchezza sociale la ricchezza mafiosa non è un valore economico: è un valore simbolico, e tutti coloro i quali lavorano su queste questioni - mi lasci dire, a cominciare dal sottosegretario Mantovano,

(lo dico sapendo il sacrilegio che compio): è una delle organizzazioni più strutturate dal punto di vista culturale, simbolico e politico che si conosca. Generale Ramponi, questo è il punto! Il fatto che un capomafia torni ad abitare un luogo che potrebbe diventare una caserma o una scuola, vale... dal Gruppo PdL).* Vale molto, ma molto di più di quanto non possa valere sul mercato quell'immobile, anche sopravvalutato. Questa è la questione. nessuno sta dicendo che qualcuno vuole agire intenzionalmente o che ci sia - neanche lontanamente è ipotizzabile - una corresponsabilità. Stiamo soltanto richiamando l'Aula del Senato a una valutazione più profonda - mi lasci dire - di questa disposizione: né più, né meno.

Signor Presidente, l'emendamento 2.37 riguarda l'istituzione di un Fondo per le crisi di mercato agricolo. Come Partito Democratico da oltre un anno abbiamo chiesto un piano straordinario per l'agricoltura. La risposta è stata il semplice ripristino delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, ma con coperture in parte virtuali e ipotetiche, alcune risorse poco più che simboliche per il credito agricolo e microproroghe per quanto riguarda gli sgravi fiscali per la previdenza. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su tale emendamento. Noi non abbiamo più parole per cercare di descrivere lo stato d'emergenza del settore agricolo. Gli agricoltori lo stanno facendo da mesi in centinaia di piazze in Italia. Allora lascio parlare i numeri, che non sono né di destra né di sinistra: i numeri evidenziano che l'*export* delle nostre produzioni agricole è in crollo, con picchi di meno 21 per cento per quanto riguarda l'ortofrutta,

Potrei parlare dell'olio d'oliva, del latte, della zootecnia, dei prodotti lattiero-caseari, a fronte di un costo di produzione che ormai ha raggiunto un più 26 per cento. In sostanza, per tutto il 2009 la maggioranza delle imprese agricole ha lavorato in perdita, e ce lo mostra in questi giorni un dato di Eurostat:

Allora, 150 milioni per far fronte all'emergenza di mercato, per scongiurare il rischio dell'uscita di produzione di molte aziende agricole, soprattutto quelle ad alto impiego di capitali e professionalità, professionalità, è il minimo di reazione di un Paese che tiene al suo settore primario. Se non c'è neppure questo, mi chiedo come continuerete a giustificare che le risorse che avevate le avete allocate diversamente; mi chiedo come direte agli agricoltori che non mettete 150 milioni ma prevedete ben 2 miliardi e mezzo in più per pagare l'ICI ai l'ICI ai contribuenti più facoltosi, misura di cui si fa fatica a vedere la finalità strategica in tempo di crisi. Quindi rivolgo un appello ai colleghi affinché ci sia almeno un provvedimento davvero anticrisi per il settore agricolo.

Signor Presidente, vorrei rivolgere un appello all'Aula perché possa riconsiderare l'emendamento 2.59 con la necessaria e dovuta attenzione.

delle tutele e delle protezioni sociali. È un argomento particolarmente attuale, se consideriamo che il ministro Sacconi proprio

sono state accolte dall'INPS 1.500. Non abbiamo bisogno di usare un'affermazione ormai consumata da parte del Governatore della Banca d'Italia, il quale ci ricorda

le mozioni approvate durante una straordinaria seduta di discussione sugli ammortizzatori sociali erano molto chiare.

«una drastica semplificazione dei tempi e delle procedure di erogazione di tutte le tipologie di ammortizzatori sociali» e «adeguate forme di sostegno a chi, specie se assunto su base temporanea o con contratti atipici, perde un lavoro

che impegnava il Governo ad avviare procedure «in favore di nuove politiche a tutela dei soggetti più deboli e in particolare di donne, giovani, famiglie, inabili

Crediamo però che il modo di procedere, le parole, la forma, che è anche sostanza - in questi giorni tanto lo sentiamo dire anche dal Capo dello Stato -, usate dall'ingegner Moretti non siano adatte a trattare le questioni del Paese.

Signor Presidente, intervengo relativamente all'elezione dei due nuovi senatori Segretari d'Aula prevista per questo pomeriggio, elezione alla quale non parteciperò, per i motivi esposti durante il dibattito sulle modifiche regolamentari. Se non ricordo male, ci è stato detto che continueremo a votare fin quando non verrà eletto un rappresentante del Gruppo che non risultò tra gli eletti

dovesse risultare finalmente un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori che il giorno dopo passa al PdL, all'UDC o al PD, cosa succede? Si ricreano altri due Segretari d'Aula, che saremo tutti riconvocati a eleggere? Questo è quello

per il prezioso lavoro che sta svolgendo per la soluzione di tutte le situazioni di crisi. In particolare, desidero evidenziare in questa sede la crisi che si è determinata per l'azienda Yamaha di Lesmo.

l'azienda dimostri, anche per la pressione che il Governo sta esercitando, di accettare la cassa integrazione.

questa condizione, invero particolare, nella quale si trovano i lavoratori della Yamaha. Il Governo, come gentilmente ha ricordato la senatrice Baio, ha convocato le parti, esercitando una legittima sollecitazione

la continuità, entro certi limiti, del rapporto di lavoro, affinché sia dato modo anche alla Regione di svolgere politiche attive di ricollocamento delle persone stesse. Purtroppo, la natura multinazionale della compagnia fa sì che il *management* italiano non abbia un'autonomia decisionale. Abbiamo rappresentato tutte le conseguenze possibili di una rigidità inaccettabile e incomprensibile,

nel nostro mercato di consumo: certo, anche noi ci troveremmo a spendere parole che inevitabilmente si rifletterebbero sulla credibilità del marchio stesso in questo mercato.

volere una soluzione che è a portata di mano, e che confido nelle prossime ore possa essere prodotta, mettendo i lavoratori nella condizione di affrontare un Natale meno drammatico: non dico sereno perché, purtroppo, né per loro, né per altri lo sarà, data l'incertezza

rende questo Natale per tanti lavoratori, costretti a salire sui tetti per difendere il loro posto di lavoro, un Natale triste. Le responsabilità sappiamo di chi sono: sono di quei banchieri a cui non importa nulla di fare la parte dei cattivi, gli stessi

il signor Lorenzo Torto, di anni 22, diversamente abile dalla nascita, che dopo numerosi tentativi falliti di ricercare un posto di lavoro presso enti pubblici e privati si è visto costretto ad interpellare il Presidente della Repubblica, il quale, a sua volta, avrebbe incaricato del caso il prefetto di Chieti affinché si interessasse presso le istituzioni. A tutt'oggi, nonostante siano trascorsi tre anni, la richiesta di aiuto non avrebbe ricevuto alcuna risposta da parte delle istituzioni. Signor Presidente, sollecito ancora una volta la risposta del Governo, perché ricordo che la legge n. 68 del 12 marzo 1999 stabilisce il diritto al lavoro per le persone diversamente abili, sia in enti pubblici che in società private, prevedendo il collocamento mirato costituito da un insieme di strumenti tecnici e di supporto volti a valutare la capacità lavorativa della singola persona disabile e ad analizzare la caratteristica di ogni posto di lavoro al fine di inserire il disabile nel posto più adatto alle sue esigenze e alle sue potenzialità. Lo chiedo,

Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, per carattere tenderei a non sollecitare le interrogazioni, perché penso che il Governo prima o poi si farà carico

confinante con Verona, ma anche con la provincia di Mantova. La Regione Veneto, in dispregio sia al piano territoriale di Verona sia ai piani territoriali confinanti, ha dato la concessione per la costruzione di

che la viabilità interromperà i flussi facili di percorrenza, con conseguente sciupio energetico e problemi ecologici. La mia interrogazione è rivolta all'intero Governo, perché riguarda sia il territorio, sia l'ambiente, sia le competenze periferiche. Il Governo, nella sua capacità ispettiva, veda se davvero, anche nella logica federalista, una Regione può prevaricare il territorio di un'altra Regione, fare in modo che gli enti locali attraverso la loro programmazione vengano superati dalle Regioni. È un'interrogazione che dallo specifico arriva al generale, perché tratta di una politica sulla quale questo Parlamento è impegnato nel voler valorizzare territorio, ambiente, ecologia ed enti locali.